Signora Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario, la discussione di questa mozione avviene in un momento particolarmente grave e doloroso per la ricerca e l'affermazione della verità e della giustizia sulle stragi nel nostro Paese. A 36 anni dalla strage di Piazza della Loggia a Brescia, lo Stato, ancora una volta, ha alzato le mani e si è dichiarato incapace di accertare la verità, di dare nomi e volti certi ai colpevoli; di descrivere, per la giustizia e per la storia, le circostanze e le intenzioni degli autori e dei mandanti dell'attentato. Ho detto "ancora una volta". È questa, infatti, una condizione ricorrente che riguarda la lunga teoria delle stragi terroristiche, delle stragi di mafia, degli omicidi e degli attentati che hanno segnato la vita civile e politica del nostro Paese. Ad ogni processo che si chiude senza colpevoli rinnoviamo la conta: la conta dei luoghi, dei morti, dei feriti nel corpo, dei feriti nell'anima e negli affetti. Molte volte abbiamo dovuto fare questa triste conta anche nella mia città, Bologna: la strage di Ustica, il treno Italicus, la bomba alla stazione, i morti del rapido 904, l'assassinio di Marco Biagi; molte volte in molte altre città. Conte, queste, che hanno attraversato un'intera generazione: quasi quarant'anni, una vita, quasi il tempo della democrazia nel nostro Paese. Ad ogni processo concluso senza colpevoli, in luogo della verità, si diffonde nuovamente la nebbia, il dubbio, l'opacità in cui il confine tra legalità ed illegalità si corrompe; in cui l'affermazione del principio democratico sembra negata dai fatti in uno Stato che, non garantendo piena libertà e sicurezza per i propri cittadini, nega il proprio fondamento e la propria funzione; in uno Stato i cui corpi e apparati troppe volte appaiono concorrere all'occultamento della verità, quando non siano direttamente coinvolti nella violazione delle regole democratiche, nella distorsione violenta della democrazia. Ci si sente male, colleghi, e mi sento male ad essere parte in questo momento di un'istituzione. Si avverte la contraddizione profonda di essere massima istanza della rappresentanza democratica e, al tempo stesso, testimoni. È una testimonianza impossibile, perché chi deve operare per garantire pari dignità, sicurezza e giustizia ai cittadini, non può essere testimone della loro negazione. Chiediamo a questo Senato che si impegni al massimo delle proprie potestà per garantire l'accertamento della verità e l'affermazione della giustizia, per Brescia come per tutti le altre stragi ed omicidi. La posta in gioco è il rispetto della vita e della dignità umana, la funzione e la dignità delle istituzioni e, da ultimo, il fondamento stesso della democrazia. Ugualmente - su questo specifico aspetto insiste la mozione che presentiamo questa mattina - è fondamentale l'impegno a garantire "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" previsto dall'articolo 3 della nostra Costituzione nei confronti delle vittime e dei loro familiari. Questo è lo spirito è lo scopo della legge n. 206 del 2004, approvata unitariamente nei due rami del Parlamento. Nelle motivazioni sottese alla sua assunzione si legge: «È in forza del legame di appartenenza alla comunità democraticamente fondata, contro cui è stata portata una vera e propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro familiari sono resi destinatari di una normativa affatto speciale, caratterizzata da istituti che postulano (...) benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali», così rendendosi il Parlamento «interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo, durante una lunga stagione che ha visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle istituzioni, soggetti aventi ruoli e responsabilità nell'ambito del sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e molti comuni cittadini». Ora, nell'applicazione di questa legge sono state riscontrate, nei sei anni dalla sua emanazione, innumerevoli difficoltà da parte degli enti previdenziali e delle articolazioni dello Stato a diverso titolo preposte al riconoscimento della condizione dei beneficiari

così come sono state escluse dai benefici quelle persone conviventi che, pur essendo parte integrante delle famiglie delle vittime, al momento dell'atto terroristico non erano legate a queste dall'istituto del matrimonio. Incertezze ed interpretazioni contraddittorie riguardano il riconoscimento del diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi - spettante ai sensi dell'articolo 3 della legge per legami parentali intervenuti dopo l'atto terroristico. Del pari si riscontrano difficoltà al riconoscimento del diritto alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, che deve essere indipendente della capacità lavorativa, che deve essere indipendente dal momento di apertura della posizione assicurativa, ovvero, per essere chiari, dal fatto che la vittima fosse o meno in condizione lavorativa nel momento in cui è rimasta vittima dell'attentato. Ancora, devono essere applicate procedure coerenti e criteri di equità ed omogeneità nel riconoscimento e nella revisione delle invalidità derivanti dagli stessi atti, nella rivalutazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali, nella restituzione degli importi relativi a versamenti fiscali e contributivi non dovuti, nel riconoscimento della decorrenza e nella liquidazione delle provvidenze. Devono, infine, essere rese coerenti le disposizioni contenute nelle diverse leggi che assimilano le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi alle vittime del dovere e della criminalità organizzata. Tutto ciò si rende necessario a fronte delle incertezze conseguenti a diversi orientamenti espressi dalle amministrazioni preposte o promananti addirittura da sentenze. Un'osservazione su questo aspetto: è impensabile ed indicibile che persone costrette per decenni al rapporto con una funzione di giustizia che non riesce ad esprimere il proprio fine con l'accertamento delle responsabilità, siano costrette a rivolgersi nuovamente ai tribunali e a frequentarli anche per veder riconosciuto pienamente il loro diritto al risarcimento ed alla solidarietà. È un orrendo contrappasso imposto alle vittime, anziché ai colpevoli. Dove si verifichi che il pieno riconoscimento dei diritti delle vittime e dei loro familiari secondo criteri di equità ed omogeneità richieda interventi normativi, la mozione impegna il Governo a un loro esame e ad una rapida assunzione e attuazione. Nella direzione fin qui tracciata ed auspicata si sono mossi diversi livelli istituzionali; alla Camera sono stati approvati ordini del giorno *bipartisan* in diverse e successive sessioni, dal 2007 fino ad oggi. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gianni Letta, in due occasioni successive nel corso di questa legislatura (precisamente nel novembre 2009 e nello scorso giugno) ha sollecitato le istituzioni e gli enti interessati a porre in atto tutte gli interventi necessari a dare piena e rapida soluzione ai problemi riscontrati, rassicurando contestualmente le associazioni delle vittime (in particolare l'AIVITER e Unione familiari vittime per stragi) che in tal senso si sarebbe operato. operato. Infine, l'ultima e superiore istanza, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della Giornata della memoria lo scorso 8 maggio ha rivolto al Governo l'invito a sciogliere i nodi che rendono ancora incerto e precario l'insieme dei diritti, pure riconosciuti per legge, a chi è sopravvissuto e ai familiari delle vittime. Da ultimo, dispositivi che chiedono al Parlamento ed alle istituzioni di impegnarsi in tal senso sono stati approvati all'unanimità, oltre che da molti enti locali e Regioni,

In questo quadro chiediamo quindi che un orientamento di giustizia, che appare condiviso da tutte le forze politiche e da diversi livelli istituzionali, non rimanga ancora una volta mera affermazione, ma si concretizzi in azioni del Governo e, laddove necessario, in interventi legislativi - sui quali anche il Gruppo del Partito Democratico è è direttamente impegnato - affinché tante sofferenze e tante difficoltà, anche economiche, non debbano prolungarsi ulteriormente, ma trovino finalmente un'adeguata risposta da parte delle istituzioni.

quanto riguarda la mozione in esame occorre dire che il sistema processuale italiano, ripensato con la riforma del 1988, è stato caratterizzato da un'attenzione specifica alle esigenze della persona offesa dal reato, riservando ad essa spazi costituiti dall'attribuzione di facoltà e di diritti in ogni stadio della procedura, al punto da dedicare alla persona offesa dal reato un intero titolo del codice di procedura penale, significativamente inserito tra quelli relativi ai soggetti del procedimento. Nonostante le intenzioni del legislatore, oggi la vittima del reato è di fatto un soggetto privo di qualsiasi rappresentatività. La vittima non è adeguatamente sostenuta in ambito giudiziario, specie in tema di supporto psicologico e di assistenza; è vulnerabile ed è fortemente esposta al rischio e ad un forte livello di sofferenza che si sviluppa in conseguenza della sua condizione di vittima. Il Consiglio europeo, con decisione del 15 e 16 ottobre 1999 assunta a Tampere, in Finlandia, ha determinato l'istituzione di norme minime per proteggere le vittime della criminalità, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e al risarcimento dei danni e con la successiva decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, viene sancito un profondo cambiamento culturale, che assegna alla vittima un ruolo più attivo e centrale nell'ambito del procedimento penale e riconosce loro diritti e bisogni, garantendone finalmente dignità e rispetto. Anche la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004, nel ripercorre il medesimo indirizzo, prevede che ciascuno Stato membro realizzi un sistema nazionale che assicuri un giusto ed adeguato risarcimento alle vittime di reati. La scarsa - o, purtroppo, nulla - percezione sociale delle vittime dei reati è il risultato di un processo complesso, ma le sue conseguenze sono purtroppo assai gravi. Occorre quindi consapevolmente considerare che ogni reato determina, nei confronti di chi lo subisce, un impatto di tipo traumatico di forza variabile, che provoca delle reazioni di diversa misura ma che certamente possono diventare invalidanti nella vita della vittima. Diviene quindi molto più difficile - talvolta impossibile - superare completamente le sofferenze psicologiche e morali indotte da un atto criminoso, senza contare i problemi materiali - primi fra tutti, quelli economici - che spesso si manifestano, contribuendo ad aggravare il cosiddetto danno secondario, determinando un clima di diffidenza e di distacco nei confronti delle istituzioni, percepite molto spesso come lontane e indifferenti, la cui manifestazione più evidente è la sfiducia nei confronti dello Stato, che finisce per rendere ancora più invisibili le vittime stesse. Subire poi un reato violento, quale un abuso sessuale, oppure la perdita di un congiunto in relazione alla commissione di un reato, rende le stesse vittime ulteriormente vulnerabili, fragili ed impotenti, con un gran bisogno di protezione e di soddisfacimento dell'azione riparatrice del danno arrecato. Occorre, all'interno del procedimento penale, ridare centralità alla vittima del reato; tale percorso giuridico dovrà essenzialmente farsi carico di una riforma dell'articolo 111 della Costituzione, offrendo alla vittima un'autonoma posizione processuale. L'istanza attuale non è più assolutamente rinviabile; dobbiamo offrire alla vittima un immediato riparo all'offesa subita, indennizzandola in maniera equa ed adeguata.

che imponeva a tutti gli Stati membri di prevedere nella rispettiva legislazione nazionale un sistema di indennizzo delle vittime dei reati violenti. Ciò muove dall'assunto riferibile alle oggettive difficoltà incontrate dalle vittime per ottenere equa riparazione al danno al danno subito in conseguenza del reato, in quanto l'autore non dispone delle risorse finanziarie necessarie, ovvero perché non sempre è possibile identificarlo, oppure perché la vittima non può sopportare il peso aggiuntivo delle spese legali riferite all'azione per il recupero delle somme deliberate nella sentenza di condanna. Avviene quindi che la vittima del reato rimanga, pur in presenza di una sentenza di risarcimento del danno, non retribuita dal punto di vista economico. con un disegno di legge, il nostro movimento, la Lega Nord, intende realizzare un percorso che - come osservato dall'Unione europea - realizzi una piena centralità processuale della vittima, prevedendo per le vittime dei crimini violenti un'assistenza di natura economica in grado di alleviarne il disagio, disagio, nei casi in cui l'autore di determinati reati non sia stato identificato, ovvero sussistano ragioni che rendano indispensabile, in assenza di altre fonti, un contributo equitativo al suo ristoro finanziario da parte dello Stato, con la previsione di un fondo di solidarietà. *(Applausi dai

A distanza di 36 anni dallo scoppio di una bomba in piazza della Loggia, avvenuto il 28 maggio del 1974, che causò otto morti e 103 feriti

dopo 17 anni di inchiesta, 2 anni di processo, 166 udienze dibattimentali, 7 giorni di camera di consiglio, 422 testi sentiti in aula e oltre 600 acquisiti tramite verbale, si è dovuto constatare che non c'era la prova della colpevolezza degli imputati, perlomeno al di là di ogni ragionevole dubbio, così come vuole il nostro codice.

purtroppo tutti - il Paese, il Governo, questo Parlamento - devono prendere atto che dopo 36 anni un evento così tragico e drammatico per la vita del nostro Paese resta senza colpevoli.

così composto vi sia un invito, una richiesta, un monito per chi è chiamato ad avere responsabilità istituzionali: fare in maniera, al di là degli schieramenti, delle valutazioni, delle discussioni, che nel nostro Paese le cose non vadano più così. Questa strage non entrerà più

e complesso. Proprio in una settimana così amara da questo punto di vista, la mozione che è stata illustrata dalla senatrice Ghedini assume ancora più significato, non solo come monito e richiesta di impegno al Governo perché si rimuovano gli ostacoli che si frappongono al completo adempimento delle disposizioni di legge,

di stragi, di fatti di terrorismo non si trovi anche nella condizione di essere abbandonato, non sufficientemente assistito, o

a chiudere una legislatura senza avere di certo messo in campo quei cambiamenti, quelle modifiche e quelle riforme che tutti auspicavamo. Però, in tema di giustizia, ricordiamo che noi siamo in un in un Paese dove dopo 36 anni una strage che ha visto la morte di otto persone e 103 feriti resta impunita e non vi è nessun colpevole.

in relazione a entrambe le mozioni, che tengono conto delle istanze formulate dall'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione, segnalate anche all'attenzione del Presidente della Repubblica in occasione della giornata dedicata alle vittime del terrorismo e delle stragi, esse indicano nella legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni, la struttura portante della materia in esame. In questi tre anni, dal 2008 al 2010, la Presidenza del Consiglio ha svolto un'attività di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione della normativa sulle vittime del terrorismo, attraverso la programmazione di ripetuti incontri, in costante scambio di informazioni anche con le associazioni delle vittime, in vista di una piena attuazione della legge n. 206 del 2004. Il risultato di questi incontri si è tradotto nell'impegno, da parte delle amministrazioni, a rendere più spedita ed efficiente l'applicazione della legge n. 206 del 2004, con riguardo agli adempimenti amministrativi e ai provvedimenti normativi. Si sottolinea, a questo riguardo, che gli elementi informativi concernenti la mozione in oggetto sono stati ottenuti dalle amministrazioni di competenza in occasione delle attività svolte dai vari gruppi di lavoro. l'interpretazione delle norme concernenti i benefici pensionistici sono stati interessati l'INPS e l'INPDAP, per l'adozione di una serie di provvedimenti interpretativi che consentissero l'estensione di alcuni benefici. Ai fini di una più spedita erogazione, l'INPS ha centralizzato le procedure per l'attribuzione dei benefici pensionistici. Inoltre, sul diritto immediato alla pensione pari all'ultima retribuzione percepita si è espresso, con parere reso nell'adunanza del 30 settembre 2009, il Consiglio di Stato, affermando che il beneficio può essere garantito e riconosciuto solo a chi risultava titolare di una posizione contributiva.

sono stati richiesti agli enti previdenziali elementi in merito alle pratiche pensionistiche giacenti e in situazioni di arretrato. l'INPDAP ha comunicato che non vi sono pratiche inevase e che il numero di prestazioni pensionistiche in pagamento è pari a 283. L'INPS ha comunicato invece a sua volta di aver ricevuto 340 domande e di averne definite 290 (50 risultano in istruttoria). Dai riscontri delle amministrazioni è comunque emerso che buona parte delle richieste delle associazioni non poteva essere accolta attraverso un'interpretazione estensiva della legislazione in vigore, ma soltanto attraverso disposizioni legislative. Non sono mancati, infatti, interventi legislativi, tra cui, da ultimo, si segnala il decreto legge n. 152 del 2009, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, che disciplina i benefìci a favore delle vittime del terrorismo. Per l'attribuzione ai superstiti delle vittime delle pensioni di reversibilità e indiretta, gli enti previdenziali e le amministrazioni competenti si sono fino a questo momento basati sui criteri ordinari, riconoscendo il diritto ai congiunti solo se conviventi e in posizione di dipendenza economica. Con l'interpretazione introdotta dal decreto-legge n. 152 del 2009, la pensione di reversibilità o indiretta potrà essere riconosciuta ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, se unici superstiti, sulla base del solo rapporto di parentela con la vittima, indipendentemente dagli altri requisiti ordinariamente richiesti, quali la convivenza e la mancanza di autosufficienza

comma 26, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha esentato dall'imposta di registro e da ogni altra imposta le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni,

stabilito un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro per gli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione. Ad alcuni benefici previsti dalla legislazione a favore delle vittime del terrorismo è stata data concreta attuazione anche attraverso la normativa di rango secondario. Mi riferisco al decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2009, n. 58, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2009, che ha innovato e semplificato le procedure dì assegnazione delle borse di studio,

che ha definito i parametri dì calcolo per la valutazione, consentendo alle Commissioni mediche ospedaliere di operare per riconoscere l'aggravamento delle invalidità. dal senatore Vallardi, come ho già detto, pone invece maggiormente l'attenzione sulle disfunzioni degli aspetti processuali. In linea con le osservazioni espresse dalla stessa mozione, ribadisco che effettivamente sono da registrare alcune disfunzioni che, più che alla normativa o alla carenza di previsioni legislative, sono da attribuire alla pratica applicazione di un tale consistente *corpus* di norme legislative e regolamentari. Con riferimento alle problematiche afferenti, però, agli aspetti processuali, si fa presente che sono allo studio dei competenti uffici i necessari approfondimenti. che, tenuto conto dell'attività svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e delle leggi approvate in questi tre anni, possa pervenirsi a un unico dispositivo che recepisca

in questi termini: «impegna il Governo a proseguire la promozione e il sostegno di ogni iniziativa volta a rimuovere ostacoli che impediscono alle vittime del terrorismo e ai loro familiari di accedere ai diritti loro riconosciuti, in base a quanto già previsto dalla legislazione vigente, onde riaffermare, mediante la piena ed attuale efficacia delle norme, i principi che sono alla base della legge 3 agosto 2004, n. 206; impegna inoltre il Governo a valutare le proposte di modifica legislativa e le osservazioni dell'AIVITER e dell'Unione familiari vittime per stragi».

Presidente: mi pare che le modifiche proposte dal Sottosegretario colgano - avevo dato atto anche io dell'azione svolta in questi due anni dal Governo - la necessità di rendere il percorso amministrativo il più coerente possibile con lo spirito della legge. In questo senso, occorre certamente che si superi la fase dei confronti e che si definisca un punto di responsabilità auspicabilmente unico, a livello dell'amministrazione centrale, tra le diverse amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali preposti, onde evitare rimandi inefficaci. Prendo positivamente atto anche della disponibilità di affrontare la valutazione di un percorso legislativo, al quale parteciperemo.

gli italiani vittime del terrorismo sono numerosi, e numerosi sono gli episodi, che non riguardano soltanto la stagione buia degli anni di piombo e la sua coda, che si estende fino al decennio appena trascorso: riguardano anche la stagione delle stragi mafiose; riguardano gli atti di terrorismo che hanno colpito i nostri connazionali, soprattutto negli ultimi anni, nelle missioni di pace all'estero. Le mozioni sulle quali siamo chiamati ad esprimerci oggi non costituiscono una semplice dichiarazione di impegno al Governo, anzitutto perché non rappresentano una richiesta come le tante che vediamo passare in quest'Aula. Esse, secondo noi, contengono l'espressione di un atto di civiltà, perché sono un nuovo, forte richiamo ai doveri dello Stato nei confronti di coloro che, incolpevoli, hanno subìto la violenza terroristica e di coloro che, a seguito di questa stessa violenza, sono stati privati degli affetti più cari. È quindi anche un gesto importante nel rispetto della memoria di tutte queste persone e dei loro familiari. C'è chi ha espresso manifestazione di vicinanza e sostegno morale, propria e di tutti noi, scrivendo la storia di molti di essi per mantenerne viva la memoria. È questa la prima forma di risarcimento civile e morale di fronte all'indifferenza nella quale sarebbero altrimenti caduti, costretti addirittura a far i conti, come purtroppo è spesso accaduto, con sentimenti di vergogna e umiliazione. La memoria, però, si deve poi tradurre in atti concreti di supporto e di assistenza, anche finanziaria. Ed è questo lo spirito che ha animato le iniziative legislative che, negli ultimi anni, hanno risposto concretamente alle necessità delle vittime e dei loro cari.

alle quali è seguita una copiosa emanazione di norme regolamentari e applicative), estendendoli anche alle vittime delle stragi terroristiche compiute sul territorio nazionale o extranazionale e ai loro familiari. Dopo diversi anni dalla emanazione di queste importanti leggi, le associazioni rappresentanti dei familiari delle vittime, soprattutto, ci segnalano - purtroppo - la presenza di ostacoli, in molti casi di natura interpretativa delle norme, che ne impediscono la effettiva e corretta applicazione.

Sì, è vero che la vecchia legge finanziaria era il luogo del cosiddetto assalto alla diligenza: il mio personale assalto alla diligenza, allora, come relatore, fu di stanziare 5 milioni di euro per equiparare le pensioni

non solo non erano in grado di risarcire le vittime, ma neppure di pagare le spese del processo che, in solido, ricadevano sui parenti delle vittime. È successo nel processo alle Brigate rosse per il primo loro eccidio, con l'uccisione di Mazzola e Giralucci a Padova nel 1974, nella vecchia sede del Movimento sociale. sociale. Quel processo mi ispirò quell'emendamento, e almeno quella piccola vergogna l'abbiamo cancellata: le spese processuali in quel caso, quando dovrebbero pagarle gli autori degli eccidi e questi per pagarle, almeno le paghi lo Stato e non ricadano sulle vittime stesse. Se, come si diceva, alla memoria devono seguire atti concreti come questo, è nostro compito oggi, in quest'Aula, fare sì che l'impegno concreto assunto dallo Stato

di impegnare il Governo stesso a provvedere con le iniziative più opportune alla rimozione di tali ostacoli, degli ulteriori ostacoli che rimangono indicatici dalle associazioni dei parenti e dei figli delle vittime, rendendo certe e semplici le procedure, al fine di pervenire all'applicazione della citata legge secondo gli originari principi ispiratori. *(IdV)*. Signora Presidente, colleghi, gli anni di piombo sono stati per il nostro Paese uno dei periodi più bui e tragici della storia repubblicana. Dalla fine degli anni Sessanta fino all'inizio degli anni Ottanta, i principi basilari della convivenza democratica sono stati messi in serio pericolo. Brutali atti di sangue hanno spezzato la vita di centinaia di civili, nonché di fedeli servitori dello Stato, come magistrati, avvocati, poliziotti e carabinieri. Su tutti gli attentati spiccano la strage di Piazza Fontana, ancora senza colpevoli, avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969, in cui rimasero uccise diciassette persone, e 1'assassinio del commissario

sono solo due delle numerose vittime di quella stagione di odio e violenza che deve rimanere ben scolpita nella nostra memoria al fine di bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di risveglio di quel fanatismo ideologico-politico che, in quegli anni, ha fatto tanti, troppi danni. L'incontro avvenuto al Quirinale il 9 maggio dello scorso anno tra la vedova Pinelli e la vedova Calabresi ha sicuramente rappresentato un evento dal forte valore simbolico. In quell'occasione, sono state superate posizioni e distanze che, per quarant'anni, si erano rivelate incolmabili ed è stato riscoperto il valore della solidarietà e il rifiuto della vendetta. La data scelta per la commemorazione delle vittime del terrorismo, il 9 maggio, appunto, è significativa. Il 9 maggio di 32 ani fa, infatti, con il ritrovamento in Via Caetani del corpo senza vita di Aldo Moro, veniva sferrato l'attacco più alto alle istituzioni. In quell'occasione, nei 54 giorni che separarono il rapimento dal ritrovamento, i tentativi di trattativa tra le istituzioni e le Brigate rosse hanno tenuto l'Italia con il fiato sospeso, fino alla drammatica, forse prevedibile, fine. Due anni dopo, il 2 agosto 1980, si chiudeva il periodo stragista e il presidente della Repubblica Pertini, in lacrime, davanti alle telecamere, definiva l'appena compiuta strage di Bologna come «l'impresa più criminale avvenuta in Italia». Strascichi di quelle stragi sono oggi però ancora presenti e la magistratura, così come le istituzioni, hanno l'obbligo di perpetrarne la memoria, di fare chiarezza e di far capire alle famiglie delle vittime che il loro sacrificio è stato per la Patria, per la democrazia e per la legalità, e che noi saremo sempre al loro fianco. Per questo motivo chiediamo al Governo un maggior impegno nella rimozione dì tutti quegli ostacoli di carattere burocratico e non solo, che impediscono l'efficace applicazione dell'impianto normativo esistente in materia, e, nello specifico, della legge 3 agosto 2004, L'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato, proprio in merito a quest'ultima previsione normativa, ha sottolineato alcune criticità. L'AIVITER si lamenta, infatti, della lenta applicazione, da parte dell'INPS e dell'INPDAP delle proprie circolari (rispettivamente la n. 98 del 2008 e la n. 30 del 2007). Tale ritardo comporta una tarda ricostituzione del quadro pensionistico previsto a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari. L'Associazione denuncia, inoltre, una difformità, sul territorio nazionale, nell'interpretazione, alle volte restrittiva, delle sopra citate circolari. Ciò comporterebbe, in presenza di requisiti pensionistici simili, trattamenti economici difformi. L'Italia dei Valori si dimostra da sempre sensibile alla tutela delle vittime degli atti terroristici e ha deciso quindi, anche in questa occasione, di ribadire il proprio impegno. Lo faremo nonostante il condannabile atteggiamento tenuto dall'AIVITER alla richiesta da parte nostra di informazioni e di collaborazione nella fase di presentazione in Aula della mozione n. 302. raggiunti con estrema difficoltà, si sono infatti dimostrati restii e non disponibili all'invio della documentazione da loro prodotta, asserendo di aver già trasmesso tali informazioni ad altri. Ciò nonostante, noi dell'Italia dei Valori abbiamo deciso di votare a favore di queste mozioni. Guardiamo all'interesse generale e ribadiamo con questo atto il nostro impegno a fianco delle persone le cui vite familiari e personali sono state dilaniate da tragici atti terroristici.

con le modifiche suggerite dallo stesso Sottosegretario. È vero, nel 2004 è stata emanata una norma

signor Sottosegretario, credo che quando il Capo dello Stato parla di nodi da sciogliere non si riferisca all'aspetto legislativo, ma a quella burocrazia, a quel groviglio che di solito c'è nella nostra burocrazia, sia ministeriale che di altri settori. Su questa burocrazia credo che il Governo potrebbe incidere con maggiore efficacia. D'altronde, tutto questo si potrebbe realizzare con una collaborazione e un dialogo maggiore

nonché delle vittime dei reati in generale. Da molti anni la legislazione del nostro Paese ha mostrato una doverosa attenzione nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con il cosiddetto «pacchetto sicurezza» è stato stabilito in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro annui delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; ciò dimostra che che il Governo e il ministro Maroni stanno lavorando seriamente, con i fatti e non con le chiacchiere, come qualcuno vuole far credere. Questi interventi, infatti, sono la dimostrazione del fatto che lo Stato ha voluto offrire un preciso segnale di sostegno, sia in termini morali che in termini economici, ogni volta che si trova a fronteggiare reati che sono diretti a minare le fondamenta dello Stato stesso. Nonostante tutti questi interventi legislativi, si riconosce tuttavia la mancanza di un totale coordinamento tra le diverse disposizioni di legge, che servirebbe a a rendere più razionale ed efficace la disciplina vigente in materia di tutela delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo e della criminalità organizzata. Al contempo, la strada per la piena applicazione e il completo riconoscimento dei diritti delle vittime del terrorismo non è ancora del tutto ultimata, ricordato anche il Capo dello Stato in occasione della giornata delle vittime del terrorismo, celebrata a Roma in data 9 maggio 2010. In questa occasione, il Governo è stato sollecitato a rimuovere gli aspetti della legge attuale che non consentono ancora una piena fruibilità e godimento dei diritti riconosciuti ai sopravissuti e ai familiari delle vittime del terrorismo. Esiste, quindi, tra gli impegni contenuti nella presente mozione, un preciso invito al Governo a proseguire il percorso avviato a sostegno delle persone vittime del terrorismo e dei loro familiari, promuovendo tutti gli interventi che abbiano lo scopo di garantire il pieno godimento dei diritti riconosciuti dalla legge

consistente. Non va dimenticato che, nel nostro ordinamento, non è prevista una normativa generale che tuteli tutte le vittime dei reati, e non soltanto quelle che abbiamo illustrato sopra. Infatti, Infatti, le leggi intervenute nel corso degli anni per garantire alle vittime di determinati reati l'intervento economico a carico dello Stato sono collegate dal fatto che il reato è sempre riconducibile a particolari categorie specificate in relazione a determinate contingenze. Si tratta cioè del terrorismo, della criminalità organizzata, delle richieste estorsive, dell'usura; situazioni nelle quali il legislatore ha ritenuto di doversi far carico delle conseguenze dannose di delitti di forte allarme sociale. Al contrario, manca una legge che sancisca nel nostro ordinamento una normativa generale sostanziale a tutela di di tutte le vittime dei reati. Pertanto, l'invito che rivolgo al Governo è di superare quei ritardi e vuoti normativi, fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno garantito, al fine di assicurare il pieno riconoscimento della cittadinanza processuale a tutte le vittime di reato come principio fondamentale dello Stato,

per cui nel nostro Paese è necessario un provvedimento specifico in favore delle vittime del terrorismo. La questione è legata

segnato da stragi di diversa matrice che ne hanno profondamente lacerato il tessuto civile e sociale, creando vittime inermi, innocenti, con famiglie private dei loro affetti più profondi che oggi chiedono giustizia. Chiedono giustizia perché è necessario provvedere nei loro confronti attraverso tutto ciò che lo Stato può fare; ma chiedono anche verità per quanto riguarda le stragi che hanno insanguinato questo Paese: stragi di matrice terroristica, stragi delle Brigate rosse (ricordiamo l'assassinio di Aldo Moro e della sua scorta; ricordiamo Ezio Tarantelli, Roberto Ruffilli, Carlo Casalegno, Walter Tobagi), stragi nere, stragi neofasciste, a partire da quella di Brescia, in merito alla quale ancora una volta non è stato possibile arrivare ad una sentenza in quei tribunali, oppure stragi come quella del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, per la quale c'è una sentenza definitiva che individua gli autori, nell'ambito di ambienti del neofascismo, con delle connivenze ben precise da parte di uomini che appartenevano agli apparati dello Stato. È questa la cosa più dura da ammettere, cioè che nel corso di questo tempo, anziché trovare tutti gli apparati dello Stato a favore delle vittime e impegnati nell'individuazione dei responsabili, spesso li si è trovati dall'altra parte. Anche per questa ragione è necessario dare attuazione a questa legge ed è necessario che questa stagione finisca e sia possibile avere finalmente verità e giustizia per queste povere vittime.

attesa da tempo, si era formata in modo parallelo ad una legislazione già esistente, che voglio richiamare non soltanto con la soddisfazione ma anche con l'emozione di chi alla formazione di quelle leggi ha partecipato, che hanno fatto sì che le vittime della mafia

con il soddisfacimento economico che si è voluto introdurre con le disposizioni richiamate dagli interventi dei colleghi e dalle proposizioni inserite nelle due mozioni. Il nostro dovere è fare in modo che, anche nella mancanza di proporzionalità, l'intervento della democrazia, di chi è eletto democraticamente, di noi che a questo punto portiamo qui quella che è una volontà popolare di solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità, possa trovare spazio e attuazione. Certo, ci sono dei problemi di difficile soluzione, come quello di discernere, chiarire, interpretare il concetto di convivenza, che poi è uno dei motivi di cui

deve risultare da un procedimento giuridico difficile e complesso. Mi dispiace che a questo punto la difficoltà, che ha sicuramente riflessi anche sulla

sono ben conscio e sicuro che l'attenzione del Governo, del sottosegretario Caliendo e della Presidenza del Consiglio, nonché l'intervento del sottosegretario Letta, le dichiarazioni e i richiami fatti dal Presidente della Repubblica faranno sì che quelle difficoltà della burocrazia vengano superate. Ciò, per fare in modo

nel voto del Parlamento la soddisfazione e la speranza, come richiamato anche negli interventi dei colleghi. Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

del documento approvato all'unanimità dalla Commissione antimafia

attribuisce alla Commissione antimafia l'onere di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alla sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive».

con il voto unanime di tutte le forze politiche in essa presenti, il cosiddetto codice di autoregolamentazione. Ovviamente non poteva essere altro che una sollecitazione incisiva ai partiti perché prestassero attenzione

situazioni collegate a fatti di reato di competenza della Commissione antimafia; si sollecitavano quindi i partiti a prendere posizione in ordine alle candidature. Era necessario questo passaggio della Commissione parlamentare antimafia, o era inutile? Purtroppo, la realtà che viviamo nel nostro Paese dimostra che gli sforzi di contrasto al crimine organizzato non sono mai sufficienti, essendosi verificata - e questo è un fatto ormai storicamente accertato tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 una mutazione del *modus* operandi delle organizzazioni criminali. dalla gestione del crimine in forma cosiddetta parassitaria (oltre che con forme autonome di criminalità nel settore dei traffici)

si è trasformata, in particolare nei primissimi anni del '90, in mafia imprenditrice, utilizzando quella immagine plastica abbastanza nota del cosiddetto tavolino a tre gambe, dove i tre protagonisti erano la politica, l'imprenditoria e la mafia. La mafia imprenditrice diventa, quindi, concorrente nel mercato, ma con mezzi diversi da quelli previsti dalle regole dello La mafia imprenditrice è la mafia che non ha bisogno del circuito bancario, perché può utilizzare enormi bacini di liquidità frutto di altre attività illecite. La mafia imprenditrice non opera in un regime di corretta concorrenza, ma altera i meccanismi di affidamento degli appalti, cambiando le offerte, aprendo le buste, colludendo con il politico. Questa realtà, confinata - e noi lo sappiamo storicamente, come fatto accertato - agli appalti gestiti dalla Regione Sicilia

comincia ad infettare altre zone e a coinvolgere la 'ndrangheta, che ancora non aveva scoperto questa nuova forma di criminalità.

ed è veramente preoccupante e allarmante ciò che ieri abbiamo appreso dalla relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, il metodo è arrivato nelle Regioni del Nord. Lo stesso metodo. La relazione della Direzione investigativa antimafia

un terreno fertile, frutto inevitabilmente di collusioni o di distrazioni particolarmente colpevoli.

politica, noi dobbiamo pertanto farci carico di questo problema prima che l'infezione diventi tumorale, che le metastasi sconvolgano l'economia del nostro Paese e che la criminalità vinca definitivamente, condizionando l'economia al punto che poi non si possa più fare a meno dell'economia mafiosa al costo di mettere in crisi quella del Paese. Non dobbiamo consentire questo. La difesa passa anche attraverso dei segnali forti. È vero che ciò che noi proponiamo va ad incidere anche su profili costituzionali - penso al diritto all'elettorato passivo - ma la politica deve avere la forza di dare delle risposte, specie

ciò deve rendere la politica responsabile. La politica deve avere anche la forza di dire: chi deve subire un processo per questi reati contestati faccia un passo indietro e, prima di impegnarsi in politica o di amministrare la cosa pubblica, aspetti che la sua posizione giuridica venga definita. Questa è una risposta che il Paese ha ha bisogno che venga data al crimine organizzato, altrimenti noi non lo fermiamo più, perché è un potere enorme che sta condizionando sempre di più la nostra economia. Lungo questa strada, chiediamo al Governo un impegno perché agevoli i percorsi di iniziativa legislativa, facendo mettere dei punti fermi nel contrasto al crimine organizzato e per la difesa dei cittadini onesti, dell'economia corretta, dell'imprenditore solerte e capace, ma anche vittima di concorrenze illecite. Difendiamo l'imprenditore onesto, difendiamo i cittadini onesti e affranchiamoli dall'abbraccio soffocante dei mafiosi e dei loro amici!

Presidente, abbiamo presentato un testo 2 perché nella fretta della presentazione era saltata la parte che richiamava esplicitamente il codice di autoregolamentazione antimafia. Lo dico per i colleghi, perché non so se il testo è stato distribuito e quindi mi sembrava opportuno

svolte. È stato un impegno gravoso e un momento assai importante di unità della Commissione antimafia, su un problema che deve essere trasversalmente condiviso.

Peraltro, non posso ignorare che, nel corso dei nostri lavori, come risulta

inseriti nel codice di autoregolamentazione.

alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Vorremmo che fosse estesa anche alle elezioni per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo. I rapporti tra mafia, politica ed economia sono fin troppo noti a tutti noi e hanno avuto risvolti estremamente

in un contesto assai difficile da districare, a distanza di anni, che sta dando vita a scenari inquietanti.

in maniera tale da non alterare, attraverso questo sistema, il quadro della concorrenza nel Paese. Non si vuole, quindi, che le regole vengano distorte.

o, comunque, di divieto di accesso alla pubblica amministrazione o a incarichi politici per chi avesse implicazione in reati di mafia o in reati che sono molto contigui: quelli contro la pubblica amministrazione.

Essi riguardano la perdita di condizione di eleggibilità o la decadenza dalla carica per soggetti che siano implicati, a questo punto, non soltanto in reati

Mi riferisco ai reati di corruzione, che spesso rappresentano quella zona contigua tra mafia, politica ed economia sulla quale dobbiamo assolutamente venire a incidere. Ovviamente, tutta la disciplina da noi prospettata, e sulla quale chiediamo l'impegno del Governo ad assumere le iniziative opportune,

nella legislazione nazionale. É evidente che non si possa creare una disparità di trattamento. Nel momento in cui noi vogliamo che siano adottati percorsi opportuni che disciplinino l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, non possiamo fare a meno di prendere in considerazione anche i percorsi analoghi in materia di elezioni al Parlamento europeo nella parte che interessa nostro Paese. Sotto questo aspetto, la nostra mozione è un po' più ampia rispetto a quella presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori, anche se ne contiene una parte,

e politici. Da qui si vuole anche un impegno del Governo, affinché coloro che assumono cariche di Governo dichiarino di non trovarsi in situazioni particolari, quali quelle di essere rinviato a giudizio, essere stato oggetto di una misura cautelare, anche non definitiva,

affinché il Governo, a sua volta, si autoregolamenti, così come dovrebbero autoregolamentarsi i partiti politici, dando trasparenza delle proprie scelte. Se su questa materia è possibile promuovere e ottenere iniziative legislative che siano ovviamente in linea con la nostra Costituzione, chiediamo a questo punto un impegno forte di tutto il Parlamento e naturalmente del Governo, che è presente. *(Applausi

«etica e politica» è un binomio che viene sempre più richiamato, giustamente e necessariamente, da parte dell'elettorato, in special modo dal nostro elettorato. Già Umberto Bossi negli anni Ottanta sollevò il problema della questione morale, unicamente denunciando che i partiti erano diventati delle macchine di potere, tant' è che negli anni '90 ci fu lo scandalo Tangentopoli, che fece scomparire quasi totalmente i vecchi partiti politici. I primi anni '90 sono gli anni in cui la Lega Nord ha evidenziato, giustamente, proprio la crisi dei partiti politici classici. II singolo politico, con il suo comportamento illecito, discredita un intero partito, peggio se sospettato di interessi mafiosi. Tanti partiti si sono dati un codice etico; per quanto ci riguarda non ne abbiamo bisogno, perché il nostro codice etico è nel DNA di chi rappresenta in Parlamento e nelle istituzioni locali. Il collante tra etica e politica è la trasparenza. Trasparenza che l'elettore, giustamente, richiede sempre più, specialmente agli eletti. L'elettore vuole sapere chi vota, ma soprattutto vuole sapere come lavora il candidato scelto una volta eletto. Abbiamo sempre messo davanti l'onestà, quella intellettuale e quella politica, in modo che i nostri elettori sappiano con chi hanno a che fare. Purtroppo continuano in questo Paese episodi di collusione politica e di malaffare, di collusione con ambienti mafiosi di politici che non hanno a cuore il loro elettorato e la loro terra. Questo è un problema che il Parlamento deve sradicare e debellare, altrimenti si rischia di gettare il politico onesto, bravo, dignitoso nel calderone generico del «sono tutti uguali: chi entra in politica diventa sporco». Sarebbe il più grande errore che si possa fare, un duplice errore: il primo, di scorrettezza e scarso riconoscimento verso coloro che fanno politica onestamente e con passione, coloro che credono che la politica sia un modo attraverso il quale contribuire alla qualità della vita dei propri cittadini. Il secondo errore è che, rimandando e rimandando, diamo l'impressione che ce ne laviamo le mani se non poniamo un freno legislativo a questo fenomeno, soprattutto in questa situazione di diffusione delle mafie sui territori.

Tale codice chiama in campo direttamente la politica e i partiti, non solo per quanto attiene al tema della legalità e dell'esercizio della democrazia, ma anche per il funzionamento degli apparati pubblici. Tutto ciò è strettamente legato anche allo sviluppo economico, com'è stato detto, alla competitività e alla modernizzazione del nostro Paese. Cercherò di motivare queste affermazioni. Da molti anni le indagini della magistratura e le inchieste giornalistiche ci dicono che si esercitano profondi condizionamenti delle rappresentanze politiche nelle pubbliche amministrazioni e che i fenomeni corruttivi nuocciono gravemente all'immagine ma anche all'economia del Paese. Tali fenomeni, solo apparentemente e in modo più vistoso, sembrano appartenere ad alcuni territori, come quelli del Mezzogiorno; in realtà siamo ormai edotti del fatto che essi colpiscono tutti i territori del nostro Paese. Il rapporto tra mafia e politica è inquietante e rischia di diventare endemico per l'Italia, di corrodere fino in fondo le pubbliche amministrazioni. Esso interpella in primo luogo la politica, il nostro essere cittadini e legislatori,

per evitare che le pubbliche amministrazioni siano manipolate e, attraverso questi passi, si sviluppino l'illegalità e la dipendenza. È evidente che è compito primario della politica fare in modo che i propri rappresentanti siano inattaccabili a tutti i livelli, soprattutto per quanto riguarda quelle tipologie di reato a cui ci riferiamo nella nostra mozione, facendo in modo che essi possano essere liberi da qualsiasi ricatto o pressione di stampo mafioso o per altri reati, così come abbiamo indicato, per esempio quelli che riguardano la corruzione dentro la pubblica amministrazione. Questa è la porta che apre ai fenomeni gravi e diffusi di infiltrazione e di degenerazione, che porta a realizzare una torsione delle regole attraverso la concessione anomala di appalti e lavori pubblici, che determina il controllo e l'indirizzo di flussi ingenti e consistenti di spesa pubblica. Così, quella che dovrebbe essere l'azione volta agli interessi della comunità, viene piegata ad interessi di gruppi criminali, talvolta collegati anche a gruppi politici. E per far questo allora i rappresentanti politici, i pubblici funzionari debbono essere all'altezza del compito ed al di sopra di ogni sospetto. Questo male oscuro che rischia di corrompere oltre che le istituzioni anche le nostre comunità, non riguarda solo alcuni territori ma tanti territori, non solo alcuni ambienti sociali ma tanti ambienti sociali e professionali. Il traffico dei voti, il condizionamento dei voti di preferenza, dove essi si esprimono, è sicuramente consistente, soprattutto in alcuni territori. Ormai le mafie e le cricche provano non solo a scegliere i candidati ma anche, talvolta, ad avere delle rappresentanze dirette per corrompere meglio gli apparati pubblici e l'azione appunto della politica. È evidente a tutti, cari colleghi, che nessuna legge e nessuna pena potranno essere sufficiente per debellare questo fenomeno se non agiamo dal punto di vista culturale, civile, politico, soprattutto sul terreno della prevenzione, con tutte le misure necessarie, e non solo quelle della repressione. A questi principi si ispira la nostra mozione. I principi invocati dall'articolo 97 della nostra Carta costituzionale sull'imparzialità e sul buon andamento della pubblica amministrazione sono principi da tenere fermi, in modo saldo, perché attraverso questi si tiene insieme una comunità, una condivisione di regole e si dà senso e autorevolezza alla delega che viene attribuita all'esercizio del mandato politico ed amministrativo. In queste ore, signora Presidente, abbiamo espresso tutti la nostra soddisfazione e il nostro plauso perché apparati dello Stato hanno raggiunto encomiabili risultati nella lotta contro le organizzazioni mafiose. Bene, ma la coerenza vuole che rafforziamo questa azione combattendo ogni giorno nella politica e nelle istituzioni affinché ci sia una traccia quotidiana nel funzionamento degli apparati pubblici, nelle nomine, nelle rappresentanze politiche, nei centri decisionali di potere, perché vi siano rappresentanti che sfuggano a sospetti o a ricatti, a pressioni di interessi poco trasparenti. Questa è la battaglia del giorno per giorno, meno eclatante ma più coerente, su cui misureremo la coerenza politica anche dei partiti e di quelli che su questo mostrano le carte in regola e vogliono assumersi le loro responsabilità.

il Gruppo del PdL non ha ritenuto di presentare una propria mozione su questa materia ma ha giudicato - per dirla con l'espressione della collega Della Monica - più che opportuna questa discussione. mi riservo, alla fine dell'intervento, di fare una proposta sull'ordine dei nostri lavori. Ma vorrei ricapitolare, partendo in particolare dalla mozione Li Gotti. Essa ha, a mio giudizio, il merito di riproporre alla nostra attenzione un documento che risale al 3 aprile 2007, la cosiddetta proposta

Le forze politiche si accingevano in quella fase a formare liste di candidati per le elezioni amministrative. Non ci furono, a differenza di questa volta, tre anni dopo, polemiche di carattere istituzionale sul principio, per noi molto importante, della leale cooperazione tra istituzioni dello Stato. antimafia, allora come oggi, chiese ai prefetti di fornire ogni utile elemento d'informazione in proprio possesso in ordine alla candidatura e all'eventuale elezione di soggetti, La proposta implicita era anche allora una sorta di autoregolamentazione, ma l'espressione è decisamente impropria per ragioni di valori costituzionali, ai quali mi auguro di non essere l'unico sensibile in quest'Aula. Quello che è certo è che allora

(non del ministro Amato, ma non certo dell'ultimo dei suoi funzionari: del capo di gabinetto, che era allora l'ex capo della Polizia, dottor Gianni De Gennaro).

dallo stesso previste». Il senatore Li Gotti, uomo esperto e competente, dovrebbe apprezzare questo slalom sciistico che, tradotto in termini più semplici, ma spero non infedeli, voleva dire che il riferimento legislativo c'è

non prestigiosi, non commendevoli, non trasparenti, per fattispecie di reato ben diverse da quelle previste dalla proposta di autoregolamentazione. Di qui - spero di non essere stato un interprete forzato dello spirito che anima le mozioni dei colleghi la mozione del senatore Li Gotti che, come dicevo prima, ha il merito di disincagliarci un pochino dalla polemica, dilagata anche su organi di stampa, con l'Associazione dei prefetti e con il prefetto Lombardi, in qualche misura con lo stesso Presidente della Commissione antimafia, senatore Pisanu. Accolto quindi questo merito di avere riportato nei termini più sobri e più rispettosi delle cose il principio di leale cooperazione tra poteri diversi dello Stato (i prefetti ed il Parlamento), senza indulgere al giacobinismo dichiaratorio del - credo - neoacquisito alla Commissione antimafia

ha detto che l'esperienza, un po' più significativa della precedente, è ancora insufficiente. Bisognerà con il tempo arrivare a disciplinare per legge Parlamento questa materia, stando attenti ai problemi costituzionali di salvaguardia del diritto all'elettorato passivo. Ecco perché non penso sia opportuno entrare nel merito delle singole richieste. Lo dico a proposito della mozione Li Gotti ma, se il ragionamento in questo caso è convincente, lo è a maggiore ragione per lo spettro, assai più largo, della della mozione della senatrice Della Monica. Colleghi, dobbiamo rispettare il Parlamento: abbiamo fra di noi la stessa sensibilità, la stessa cultura dell'antimafia?

ha detto di non aver nulla da vergognarsi della sua attività professionale. Però, mi consenta l'avvocato Li Gotti, rispetto a certo suo "savianismo" e non entro nel merito delle considerazioni espresse dai colleghi della Lega, perché il ministro Maroni ha risposto alla grande proprio nella giornata di ieri - non vi sembra vile e ingeneroso far apparire il senatore Miglio come un razzista? Sono stato in questa Aula sempre all'opposizione del senatore Miglio fra il 1992 e il 1994, le bocciature che mi ha inflitto ai concorsi universitari, ma è sguaiato rubricarlo senza possibilità di risposta e affidare la sua memoria a una costellazione fuori contesto di sue affermazioni. Quindi, colleghi dell'Italia dei Valori, atteniamoci al rango dei valori penultimi, e nei valori penultimi non può non esserci quello della Costituzione. Non si può prescindere dai testi costituzionali quando si legifera in questa materia. La mia proposta è pertanto di non votare nella seduta di oggi

Colleghi e amici, sono questioni più che mai all'ordine del giorno, se questa legislatura avrà un futuro. Nella Commissione affari costituzionali c'è il cosiddetto codice delle autonomie: tutti, o quasi tutti, i punti della mozione Li Gotti possono essere discussi, ma farei torto a questa Aula e a me stesso se rinunziassi in qualunque dispositivo su questa materia ad un esplicito richiamo al rispetto dei principi, dei valori, se me lo consentite, previsti nel testo costituzionale. antimafia, credo sia opportuno - e il senatore Pisanu intende convocarla - dare un chiarimento su questo ping pong con i prefetti, per considerarlo chiuso, anche grazie alle mozioni e a come sono state incardinate oggi, magari tenendo conto di altre novità che ci sono state su questo fronte. Sia gloria alla cattura del camorrista ma, venendo a sodalizi di rango superiore, ho l'impressione che finalmente, per la parola di un gentiluomo quale il professor Conso, il calvario che da molti anni subisce quella nitida figura di soldato e cittadino del generale Mori

a proporre quella formulazione per me indispensabile: il richiamo del testo costituzionale, non nel dettaglio, ma sul piano di quelli che ho chiamato i valori penultimi.

Presidente, in un accordo informale con i colleghi Capigruppo, al fine di trovare una mozione condivisa su un tema tanto delicato, delicato, il Gruppo dell'Italia dei Valori è dell'avviso di trovare un approfondimento extra Aula in modo che torni in questa sede un testo condiviso, che possa essere votato possibilmente in coda al voto finale

Presidente, noi non siamo contrari al rinvio del voto finale, ma vorremmo capire meglio qual è l'obiettivo della sospensione, perché stiamo facendo un dibattito che, al di là del merito, segnala una criticità del sistema politico partitico. infatti, siamo costretti a discutere di tali questioni, è perché stiamo partendo dal presupposto dell'incapacità dei partiti e di chi fa selezione di classe dirigente di esprimere un personale politico selezionato sulla base della responsabilità e dell'etica pubblica. Forse è questo il vero approfondimento che dovremmo fare e non credo che a tal fine possa bastare il rinvio del voto delle mozioni.

norme che riguardano l'articolo 58 del testo unico degli enti locali e, altresì, tutta una serie di reati che determinano l'incandidabilità.

e principi affermati nella nostra Costituzione. Lo stesso disegno di legge disciplina le cause di non eleggibilità alla carica di deputato e di senatore

dal senatore Li Gotti attiene esclusivamente alle elezioni degli enti locali e dunque all'articolo 58 del testo unico,

siamo proprio convinti che, di fronte a queste motivazioni, che tutti conoscono per l'esperienza maturata da ciascuno di noi, basta questo per rendere ineleggibile

dell'ipotesi che dopo due condanne, in primo grado e in appello, non vi sia possibilità di essere eletti, ma siamo proprio convinti che il decreto di rinvio a giudizio non incida

la nostra vita, il nostro modo di operare, l'articolo 27 della Costituzione, l'ordinamento penitenziario e tutto il resto? Se diciamo che vi è un'ipotesi di esclusione permanente,

di risollevarsi, di abbandonare un sistema di vita, di ricostituire un sistema di vita legale e lecito. Come possiamo dire «in eterno»?

che è ben diverso. Una cosa sono i problemi di incandidabilità e ineleggibilità, altro è quello che attiene alla possibilità di scegliere tra coloro che devono avere incarichi o contratti. o contratti. Ho chiesto di intervenire perché questo spazio deliberante, prima di votare la mozione, possa consentire una riflessione seria su questi aspetti:

nel testo come viene proposto, nelle disposizioni, sono un po' traditi nei due aspetti fondamentali che mi trovano un po' preoccupato: il decreto di rinvio a giudizio e la perpetuità delle cause di incandidabilità od ineleggibilità. Mi sembra un qualcosa di talmente forte da negare i valori alla base di uno Stato democratico.

sull'apertura della sessione di bilancio.

La prima mozione a firma della senatrice Della Monica ed altri aveva un contenuto - a mio parere - assolutamente condivisibile, perché faceva riferimento costante alle condizioni di ineleggibilità, oggi ancora più precisate in ordine alle condanne definitive.

Ora abbiamo il problema (come è ovvio), nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, di trovare tutti gli strumenti necessari e sufficienti per frenare questo fenomeno che ci invade. Ha ragione il senatore Li Gotti quando afferma che la capacità di uniformarsi, di nascondersi e riciclarsi di questa forma di organizzazione ha bisogno di una costante attenzione.

Dal punto di vista sostanziale, basti pensare alla creazione del concorso esterno in associazione mafiosa, che è tipico di detta forma di criminalità, ma che ‑ per esempio ‑ non esiste nelle associazioni criminali di altra natura, quelle cosiddette semplici. Anche dal punto di vista processuale dell'esecuzione, abbiamo una soluzione di doppio binario: doppio binario a cui ci hanno obbligato, evidentemente, le associazioni mafiose e camorristiche di questo stampo. Lo Stato, infatti, non poteva non rispondere se non con strumenti che che imboccassero un binario diverso da quello su cui correva un treno che le associazioni mafiose facevano costantemente deragliare. Quindi, abbiamo creato un doppio binario blindato per le associazioni criminose, e mi sembra assolutamente giusto.

Non sono d'accordo con il senatore Compagna quando afferma che non bisogna entrare nel merito dei contenuti, perché certe proposte sono veramente degne di attenzione. Il decreto che dispone il giudizio, diversamente da quanto detto dal rappresentante del Governo, qualche volta è motivato,

Ed allora abbiamo l'iniziativa del pubblico ministero, o del pubblico ministero e del giudice delle indagini preliminari, che configurerebbe di per sé la ineleggibilità o la incandidabilità. A me sembra veramente eccessivo, come mi sembra eccessivo dare la incandidabilità come *capitis deminutio* - che si vorrebbe come *maxima* perché perpetua **-** a carico di chi sia stato condannato in primo grado.

alla presunzione d'innocenza nei confronti di chiunque fino alla sentenza definitiva. Era una presunzione di non colpevolezza per la cautela che aveva dettato il legislatore costituzionale, che diventa presunzione di innocenza per via del recepimento nel nostro ordinamento costituzionale dei principi dei diritti europei, che sono stati ribaditi più volte. Ecco, questo è il punto. L'entusiasmo che certamente deve sorreggere le iniziative legislative nei confronti di questi farabutti altro aggettivo o sostantivo che possa descrivere in realtà la criminalità organizzata di stampo mafioso, perché quello che fanno va al di là dell'immaginabile, dell'umano, per certi aspetti, quando si tratta

il primo testo della mozione Della Monica l'avrei votato, assolutamente,

il principio di non colpevolezza o di innocenza fino a sentenza definitiva non possiamo dimenticarlo mai.

voglio iniziare ad illustrare questa mozione (che è stata sottoscritta da moltissimi colleghi di quasi tutti i Gruppi politici presenti all'interno del Senato) riportando le parole di uno dei maggiori studiosi della materia e psicoanalisti (Carl Gustav Jung), il quale diceva che «la depressione è una signora in nero, quando appare non bisogna scacciarla, ma invitarla alla nostra tavola per ascoltare cosa ci dice». di parole suggestive e intriganti (se vogliamo), ma anche, purtroppo, molto, ma molto attuali. Le parole del grande psicanalista invitano all'ascolto di chi soffre silenziosamente e vive una condizione di costante paura e che, per questo, merita la giusta attenzione e la predisposizione di un'efficace rete di soccorso ramificata a tutti i livelli: sociale, medico e istituzionale. merita attenzione e dobbiamo farla sedere alla nostra tavola. La depressione è un male oscuro, silenzioso, che ormai affligge in modo preponderante la nostra società. Viene definito il «male dell'anima», e nessuno ne è immune, anche se le donne sono quelle maggiormente colpite: il dato allarmante in nostro possesso è quello secondo cui le donne afflitte da depressione La scienza la riconosce come una malattia curabile, una patologia dell'umore contro la quale è ormai improcrastinabile un intervento deciso e risolutivo da parte delle istituzioni affinché questo terribile male sia inserito e trattato come una priorità Siamo di fronte ad una malattia, una malattia subdola, che, nonostante i piccoli campanelli di allarme (purtroppo sono piccoli, impercettibili difficili da cogliere e riconoscere), si insinua nella vita delle persone, soprattutto delle donne, rendendole schiave all'interno delle mura domestiche, sorde e cieche nei confronti del mondo, delle gioie e della speranza. Ignorare questa malattia e questi sentimenti vuol dire rifiutarsi di prendersi carico del benessere delle persone, delle donne, dei loro figli e delle loro famiglie. Per questo oggi è quanto mai necessario e fondamentale sottolineare che la depressione è una patologia curabile: è una malattia e, come tale, è curabile. Noi dobbiamo garantire questa cura e siamo qui oggi per questo. per questo. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, tra 20 anni questo «male oscuro» colpirà più di qualsiasi altra malattia. Nel 2020 sarà la seconda causa di disabilità nel mondo e per le società diventerà l'onere sanitario più pesante, da un punto di vista sia economico che sociologico. In Italia si dice che il 18 per cento della popolazione abbia sofferto di una malattia a livello mentale (più che di una malattia, di un disagio): si parla di 17 milioni di persone e il 10 per cento di esse

Indro Montanelli ricordava che la depressione «è una malattia democratica: colpisce tutti» e molto più di tutte le altre malattie. È una malattia che colpisce in modo indifferenziato dal punto di vista sociale e geografico, nonché in relazione in relazione all'età. Il crescente onere sociale che deriva da questa malattia democratica sarà un problema di vaste proporzioni per i Paesi in via di sviluppo, che hanno a disposizione delle risorse scarsissime da destinare alle malattie mentali. I dati sono impressionanti: circa la metà delle patologie mentali viene avvertita prima dei 14 anni; e si calcola che il 20 per cento della popolazione minorile - ovvero bambini e adolescenti - abbia patologie legate alla salute mentale, o comunque problemi correlati. La gran parte delle Nazioni a basso reddito ha soltanto uno psichiatra infantile per 1 o addirittura 4 milioni di abitanti (è un dato agghiacciante). I suicidi ogni anno sono 800.000, concentrati per cento nelle Nazioni più povere; oltre la metà dei suicidi avviene tra i 15 e i 44 anni. Si tratta di un male lasciatemi usare questo termine - e distruttivo, che presenta un insieme di sintomi di natura cognitiva, comportamentale, somatica ed affettiva, che compromette l'umore, in alcuni casi in modo lieve, mentre in altri in modo molto più severo, riducendo le abilità e le capacità di adattarsi alla vita sociale; nel peggiore dei casi, purtroppo, conduce anche alla morte. La persona depressa, se non correttamente diagnosticata e curata, vede compromessa la sua personalità, il suo modo di ragionare, di pensare, di agire e di percepire se stessa e il mondo esterno. Esistono però altri fattori

che circonda le persone depresse. Già Sofocle sosteneva che «per chi ha paura, tutto scricchiola». tutto scricchiola». Ed oggi è più che mai vero. Le difficoltà economiche e di accesso alle cure psicologiche tramite il Servizio sanitario nazionale non fanno che alimentare questa paura, questa vergogna di percepirsi diverso, buttandosi alle spalle il problema con un semplice «passerà».

oltre 450 milioni di persone, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, soffrono di disturbi mentali, eppure, la gran parte delle società in via di sviluppo spende meno del 2 per cento dei bilanci nazionali per i problemi legati ai disturbi

il loro utilizzo è funzionale solo se combinato ad un efficace supporto psicologico, medico e familiare. È questo rapporto, questa rete di sostegno che deve essere offerta dalle istituzioni e dal Servizio sanitario nazionale. Come emerge da un'indagine che è stata compiuta dall'Osservatorio nazionale sulla salute delle donne, sono proprio le donne ad essere più colpite (6 su 10),

l'urlo per fare entrare in quest'Aula e in tutte le istituzioni la voce invisibile di tutte le persone che fanno fatica a vivere, a gioire e ad amare perché sono depresse. Quindi, la mozione vuole raccogliere questo urlo disperato di chi non ha più parole, affinché questo grido di aiuto possa entrare nelle istituzioni e possa far sì che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico di loro. Mutuando l'espressione di Jung, concludo ricordando che abbiamo fatto entrare in quest'Aula la «signora in nero» per ascoltarla,

ma anche che tutti i livelli sociali devono essere coinvolti con una prioritaria e indispensabile conoscenza della problematica. Vi sono depressioni legate a eventi della vita: quali i problemi del lavoro, la separazione, le perdite, le malattie. Depressioni su base fisica, connesse a disfunzioni del metabolismo, degli ormoni o ad altre cause. Si pensi alle depressioni *post partum*, a quelle da climaterio e a quelle stagionali, le cui cause sono biochimiche. Colpisce a tutte l'età, e maggiormente le donne. Si stima che una persona su quattro, nell'arco della vita, ne abbia sofferto. In Italia l'incidenza delle forme più gravi si aggira intorno al 4-5 per cento della popolazione, mentre se allarghiamo la valutazione a tutte le forme si arriva anche al 10-12 per cento. Il nodo del problema è che spesso la depressione non viene riconosciuta. Molte forme non compaiono come noi siamo abituate a pensarle, ossia con manifestazioni di tristezza, ma con una sensazione di stanchezza, di affaticamento, di dolori, disturbi che fanno pensare, a volte, soltanto a qualcosa di carattere fisico. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il 90 per cento di tutte le persone depresse non sono riconosciute come tali e, quindi, troppe volte si impedisce alla depressione di essere trattata come una malattia a tutti gli effetti. Le ragioni possono essere molteplici. La prima è la mancanza di conoscenza del fenomeno e, in secondo luogo, vi è un senso di vergogna e di disagio. Solitamente, chi ne soffre si chiude nel silenzio e pensa che non si possa fare nulla o che, comunque, tutto dipenda da una questione di volontà. Atteggiamento ma purtroppo la depressione comincia proprio laddove la volontà finisce. Non c'è infatti peggior cosa che dire a un depresso: «Dai, fai uno sforzo». La depressione comincia proprio perché finiscono le energie. Stiamo attraversando, tra l'altro, una crisi economica importante, questo è noto, una crisi che direttamente, ma anche indirettamente, colpisce tutti, nel lavoro e nella famiglia, e le donne soprattutto. Quindi, viene a crearsi un terreno sempre più fertile perché possano verificarsi episodi di depressione. Queste condizioni si creano perché alcuni punti di sicuro riferimento vengono a mancare e quindi la psiche e lo stato fisico di tanti, e soprattutto delle donne, non reggono a tutto e perciò perdono le proprie difese naturali. Quanto ho appena detto è proprio una breve sintesi di studi scientifici che mi fanno tornare alla considerazione iniziale per cui la depressione è una malattia sociale. Allora occorre intervenire così come, peraltro, è richiamato dalla mozione, a tutti i livelli. Occorre che le strutture sanitarie siano dotate di quelle risorse tali da consentire un approccio a questa malattia, che talvolta può essere devastante, come ci insegnano gravi fatti di cronaca, anche recente. Occorre, quindi, intervenire preventivamente con un'adeguata e capillare informazione, con un rafforzamento della rete assistenziale sul territorio, potenziare gli ambulatori con il supporto degli psicologi. I farmaci fanno sicuramente moltissimo, ma da soli non bastano. Quindi, è importante lo spirito *bipartisan* che ha animato la presentazione di questa mozione, che, a mio giudizio, non è soltanto un atto politico ma è un atto umano. E dietro tutti i numeri e alle percentuali ci sono dei nomi e dei volti che non dobbiamo assolutamente dimenticare.

quale connotante una sindrome psichiatrica, è stato introdotto solo negli anni Venti dallo psichiatra tedesco Adolf Meyer. Nella depressione, intesa come disturbo di rilievo clinico, il sentimento del semplice «sentirsi giù» è soltanto uno dei diversi sintomi che caratterizzano il quadro clinico e lo stato generale, che è assolutamente sproporzionato rispetto a qualsiasi causa esterna che possa averlo provocato. quindi, non ci si riferisce ad una patologia univoca, ma a una serie di disturbi, distinti tra loro, che presentano però alcune caratteristiche comuni. è già stato rilevato, l'Organizzazione mondiale della sanità stima che nel 2020 la depressione sarà una delle patologie maggiormente invalidanti al mondo, per la precisione la seconda in ordine di importanza dopo le malattie cardiovascolari. La diffusione della depressione è in continuo aumento e già oggi colpisce circa 5 milioni di persone in Italia e oltre 60 milioni in tutta Europa. un problema serio, che coinvolge famiglie e mondo del lavoro, e non di facile soluzione: una persona depressa su tre lo è ancora dopo un anno, una su dieci deve continuare la terapia dopo cinque dal primo episodio, oltre la metà avrà una ricaduta nell'arco della sua esistenza. Eppure, la gran parte delle società, soprattutto quelle in via di sviluppo, spende meno del 2 per cento dei bilanci nazionali per i problemi legati all'instabilità mentale. I dati dell'OMS rivelano che attualmente oltre 450 milioni di persone soffrono soffrono di disordini mentali, la gran parte proprio nei Paesi in via di sviluppo. E il crescente onere sociale sarà un problema particolare per questi Paesi, che dispongono di scarse risorse da destinare alle malattie mentali. I dati sono impressionanti: circa la metà delle patologie mentali viene avvertita prima dei quattordici anni e si calcola che il 20 per cento della popolazione minorile mondiale (bambini e adolescenti) abbia patologie legate alla salute mentale o comunque problemi correlati. La gran parte delle Nazioni a basso o medio reddito ha soltanto uno psichiatra infantile ogni 1-4 milioni di abitanti. I dati ci dicono che di fatto le Nazioni più povere hanno un maggior numero di depressi rispetto a quelle più ricche e che tra i poveri delle Nazioni più agiate si registra un'alta incidenza di depressione rispetto a chi ha migliori condizioni economiche nella stessa Nazione. Il professore Martin Pince, docente di epidemiologia psichiatrica al King's College di Londra, ha provato a calcolare quanto costa, in termini di costi sociali, una persona depressa. «In primo luogo bisogna calcolare la perdita di produttività perché le persone con una depressione seria trovano con maggiore difficoltà impiego e difficilmente se lo mantengono. A questo va aggiunto, almeno nelle Nazioni più avanzate, il costo degli ammortizzatori sociali. Tutti questi costi sommati ammontano in Gran Bretagna» - dove il professore ha esaminato il fenomeno - a circa 12 miliardi di sterline l'anno, circa l'1 per cento del prodotto nazionale lordo, che è davvero una somma enorme». Considerato dunque il peso sociale della depressione, che è destinato a crescere nei prossimi anni, l'OMS sostiene che va cambiato l'atteggiamento nei confronti della malattia mentale: «La depressione è una malattia esattamente come tutte le altre patologie e la gente che ne soffre ha il diritto di ricevere cura e terapia corrette, allo stesso modo che per le altre patologie sanitarie». Abbiamo visto come la depressione interessi attualmente il 10 per cento della popolazione italiana, circa 6 milioni di persone, ma ci sono anche tanti malati non diagnosticati. Ciò significa che un italiano su quattro è a rischio. dunque, essere definita la malattia di questo secolo. La gravità del fenomeno si riflette in primo luogo sulla vita delle famiglie dei malati, proprio perché la malattia incide pesantemente

Ci sono 5 milioni di italiani in terapia farmacologica, con i conseguenti costi per il sistema sanitario nazionale, ma la parte preponderante dei costi economici e sociali per il sistema è quella che proviene dalle giornate di lavoro perse, dal pensionamento anzitempo e dalle morti per suicidio. La malattia è, dunque, da considerarsi una malattia sociale e che riguarda l'intera collettività anche da un punto di vista economico. Suicidi e perdite di lavoro legate alla malattia della depressione valgono quanto una manovra di stimolo fiscale: senza il freno di questi due fattori, per esempio, il PIL giapponese di quest'anno riceverebbe una spinta addizionale di 0,4 punti, ovvero di 1.700 miliardi di yen (più di 16 miliardi di euro). Quanto al 2009, il costo calcolabile per l'economia nipponica è ammontato a quasi 2.700 miliardi di yen (25,5 miliardi di euro). Questo quadro preoccupa ancora di più alla luce della situazione economica e sociale internazionale e che il nostro Paese sta attraversando attualmente. Infatti, le prospettive almeno per i prossimi anni non sono rosee e occorrerà molto tempo prima che si riesca a tornare a livelli di reddito e di occupazione precedente la crisi Ed è soprattutto l'aumento della disoccupazione registrato nell'ultimo anno e mezzo, che non si arresterà probabilmente a breve, a preoccupare, visto che la perdita del lavoro è una delle cause principali di caduta nella depressione o di aggravamento della malattia nei casi latenti. Quindi, depressione e ansia sono le principali cause di assenza prolungata dal posto di lavoro, ridotta capacità lavorativa e prepensionamento. Il costo sociale è pari a quello sostenuto per il cancro e per le patologie cardiovascolari. Il costo sociale delle malattie mentali in Europa incide sul 3-4 per cento del PlL, secondo quanto dice una indagine condotta nel 2009 dalla Commissione salute del Dipartimento per le pari opportunità. La scarsa accettazione del prossimo nei confronti delle persone depresse e la tendenza a non chiedere aiuto, arrivando fino a nascondere, sottovalutare o negare lo stato depressivo, rendono molo difficile intervenire sulla malattia in modo preventivo. Da un recente convegno è stato lanciato l'appello a parlare liberamente della propria malattia, a non vergognarsi, ad uscire dall'isolamento: e al pari di qualsiasi altra malattia, prima ci si rivolge ad uno specialista e prima si riesce a curarla. Da un recente studio, sempre condotto dalla Commissione salute del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio su disturbi della stima, ansia, depressione ed altre patologie psichiatriche emerge che il 18 per cento della popolazione ha sofferto nel corso della vita di malattie mentali cento nell'ultimo anno. Tra queste, la depressione è risultata la malattia più comune. Sembra che il 10 per cento degli italiani ne ha sofferto nel corso della vita ed il 3 per cento nell'ultimo anno. Un fenomeno che risulta molto diffuso nelle donne e tra coloro che vivono nelle Regioni del Sud. Altro dato emerso dallo studio è che il 53 per cento degli italiani hanno avuto un contatto diretto con persone che hanno sofferto di ansia e depressione. da tutto questo è facile vedere come il fenomeno riguarda tutta la nostra società e come sia importante la mozione che oggi discutiamo e che è stata condivisa I rimedi contro la depressione sono soprattutto di carattere farmacologico e psicoterapeutico. I rimedi del primo tipo funzionano nella maggior parte dei casi. I rimedi del secondo tipo funzionano da soli solo in una casistica specifica e circoscritta: di consueto forniscono un accompagnamento alle cure farmacologiche per rafforzarne l'efficacia. Oggi si fa già molto, ma ci sono ampi spazi di miglioramento delle politiche di assistenza ai malati di depressione. Quindi per migliorare le iniziative e per fronteggiare l'emergenza bisogna considerare soprattutto due cose: innanzitutto il fatto che l'estensione del fenomeno è ancora più grave di quanto possa sembrare guardando a tutti i numeri citati nel corso del mio intervento, perché i numeri stessi descrivono solo parzialmente la situazione. Infatti, bisogna considerare che circa il 50 per cento dei casi non viene nemmeno diagnosticato, con la conseguenza che molti malati non sanno di esserlo, fino a concludere la propria vita con quegli episodi gravi e tristi che spesso leggiamo sulla cronaca. Un altro importante aspetto da considerare è la coesistenza della depressione con altri tipi di malattie. È vero infatti che in circa la metà dei casi la depressione si associa ad altre patologie gravi di natura fisiologica, probabilmente anche perché correlata a queste ultime. Parliamo di chi ha subito un infarto o un *ictus*, soffre di diabete o di ipertensione, o peggio è ammalato di cancro. Evidentemente, queste situazioni rendono ancora più palese il bisogno di queste persone di un sostegno efficace e concreto da parte del sistema pubblico. Va inoltre ricordato che è frequente, nella società contemporanea, un giudizio morale nei casi di malattie mentali e, soprattutto nel caso della depressione, un giudizio che porta a condannare, ad esempio, la "svogliatezza" della persona sofferente e ad esortarla a reagire, in nome di una richiesta di efficienza costante del corpo e della mente e di un perenne buonumore, seppur apparente. Come conseguenza di ciò, è la persona stessa che arriva a giudicarsi per il suo malessere e per le sue incapacità. Spesso infatti la poca stima, la paura e la sfiducia verso sé stessi ed il futuro sono accompagnati da giudizi severi per se stessi, per la propria inefficienza rispetto agli altri e agli standard sociali comunemente condivisi: questo porta ad un ulteriore abbattimento e ad un aggravamento della malattia. Il rischio è quello di restare nell'ombra, di nascondersi e trascurare un disturbo che invece, se ben affrontato, può essere risolto. È quindi importante che si parli di una politica di generale sensibilizzazione al fenomeno, di miglioramento delle strutture preposte alla diagnosi ed al supporto psicologico, anche attraverso l'aggiornamento di merito dei medici di medicina generale. Sono questi alcuni dei punti sui quali intervenire che sono previsti dalla mozione e che tutti noi crediamo debbano essere portati nella

*(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, abbiamo sottoscritto convintamente la mozione oggi in discussione: infatti condividiamo l'opinione che sia necessario mantenere l'attenzione su una malattia grave come la depressione la quale, com'è stato ricordato, costituisce la quarta causa di invalidità nel mondo. Ed è ancora più necessario, a mio avviso, in un momento in cui i fattori di rischio ambientale sembrano aggravarsi in conseguenza della generale incertezza sociale ed economica, che in questi ultimi anni purtroppo si è maggiormente sviluppata ed è spesso il lavoro una delle cause scatenanti il problema. È vero che le ricerche ci dicono che se lo stato di benessere personale può essere compromesso da ritmi di lavoro particolarmente intensi e tali da occupare la maggior parte del tempo; tuttavia, è difficile che questi fattori possano dar luogo allo sviluppo di una vera e propria depressione. Le stesse ricerche sottolineano altresì come sia più importante la qualità dell'attività svolta, vale a dire il modo in cui si lavora o si studia, e soprattutto le condizioni in cui tali attività sono svolte. I principali fattori di rischio individuati sono la mancanza di gratificazione e valorizzazione personale; un ambiente lavorativo caratterizzato da situazioni di conflitto, in cui il soggetto non riesce a trovare vie d'uscita o possibili soluzioni; un'errata organizzazione dei ritmi di lavoro, che porta il soggetto a ridurre progressivamente, fino ad annullarli, i propri spazi di libertà;

innegabile come, al di là dell'aspetto puramente economico consistente nella possibilità di mantenere se stessi e la propria famiglia, il lavoro sia anche uno strumento di realizzazione e gratificazione personale, di valorizzazione delle proprie capacità, di opportunità di sviluppare rapporti personali con gli altri e di mettersi a confronto con essi. Tutti gli studi concordano nell'individuare il fatto che un lavoro stabilizzato può contribuire in modo efficace a ridurre i rischi di depressione, mentre le persone che non lavorano sono più dei lavoratori a rischio di depressione. Sappiamo inoltre che la depressione crea un circolo vizioso, compromettendo in modo serio la capacità lavorativa della persona colpita: spesso la persona arriva al punto di dover addirittura smettere del tutto di lavorare, almeno per un certo periodo. Sappiamo anche che la depressione è una patologia curabile: se viene riconosciuta e la persona viene aiutata in modo opportuno essa può riguadagnare le normali condizioni di lavoro, evitando così inutili sofferenze e infelicità. Per questo è importante, come recita il primo degli impegni di questa mozione, sensibilizzare in tal senso la popolazione. I colleghi di lavoro, il più delle volte, non sono in grado di notare se uno di loro sta soffrendo di depressione ed è sempre molto difficile per tanti motivi affrontare questo argomento. Molte persone, infatti, hanno paura di parlare del loro disagio depressivo poiché temono che possa mettere in pericolo, in modi diversi, il proprio lavoro. È proprio in simili situazioni che diventa importante la conoscenza e la sensibilizzazione sull'argomento, per far sì che venga affrontato in modo adeguato, confidenziale, nel rispetto totale di chi soffre, e ciò, non solo dagli addetti ai lavori, come il consulente sanitario e il medico di famiglia, ma di tutti, perché ogni persona e ogni sua sofferenza meritano rispetto assoluto e aiuto da parte di tutti. Per la persona colpita, il primo e maggiore aiuto è sapere che non si è soli. Naturalmente è fondamentale che sia il sistema sanitario a fornire il supporto specialistico per la cura, a partire dai medici di base, che sono il pezzo del sistema sanitario più vicino ai cittadini e che con i propri pazienti hanno un rapporto più stretto. In tal senso, la formazione dei medici di base attraverso la formazione di corsi di aggiornamento sulla depressione potrà costituire un valido e vero aiuto per tutti coloro che desiderano farsi aiutare. I medici di base devono essere tuttavia solo il primo anello di quella rete di ambulatori e centri già oggi esistente, ma che va potenziata e estesa uniformemente su tutto il territorio nazionale e che deve vedere affiancato l'aspetto prettamente medico alla disponibilità del supporto psicologico, come necessaria integrazione della terapia farmacologica. Certamente deve essere assicurata la possibilità di accesso a farmaci specifici e innovativi, specialmente a chi molto spesso non può permetterseli, ma ribadiamo: il primo e più importante supporto per i cittadini cittadini colpiti da questa grave patologia è il sapere che ne possono uscire e che non saranno mai lasciati soli dalla collettività.

questa mattina siamo qui ad esporre le nostre ragioni e le nostre richieste, ben illustrate nella mozione condivisa da tutti i Gruppi parlamentari. La Lega Nord, quindi, condivide in pieno tutte le premesse e le considerazioni

spesso si presenta con sintomi lievi che però, se la donna si trova in condizioni di solitudine psico-affettiva, possono assumere connotazioni più gravi e devastanti per la donna stessa e per il neonato, soprattutto nella realtà sociale odierna, prevalentemente costituita da famiglie mononucleari, dove vengono a mancare la complicità e il supporto delle diverse figure femminili familiari. Non dimentichiamoci poi che anni fa era molto valorizzata nelle comunità locali la figura della levatrice, dell'ostetrica che anche dopo il parto si occupava della puerpera, oltre che della cura del neonato. Proprio attraverso questo interagire la depressione postparto assumeva contorni facilmente gestibili e superabili, perché anche l'ostetrica, oltre alle donne della famiglia, contribuiva, attraverso il dialogo ed il suo supporto professionale, a ridimensionare le preoccupazioni, ricollocando nel giusto ambito le ansie della mamma nei confronti della grande responsabilità genitoriale cui è chiamata dopo l'evento della nascita. Negli ultimi mesi la cronaca ci ha raccontato troppo spesso di neonati uccisi dalle mamme, di mamme che si sono suicidate dopo aver ucciso il loro figlio: certamente, alla causa principe di questi eventi, riconducibile al rifiuto o al senso di inadeguatezza nei confronti della maternità, s'intreccia la depressione postparto. Per questo motivo chiedo ai colleghi firmatari della mozione di condividere la richiesta del Gruppo della Lega Nord ed aggiungere al dispositivo un ulteriore impegno, cioè quello di accompagnare con servizi psico-sociali appropriati le puerpere nei casi in cui si riscontrassero anche forme lievi di depressione postparto. Se questo contribuisse a salvare la vita anche di un solo neonato, anche di una sola puerpera, avremmo tutti colto nel segno. Signor Presidente, nel dire che concordo con il contenuto e con l'importanza della mozione presentata dalla senatrice Baio e sottoscritta da moltissimi

una malattia con incidenza sempre maggiore e sempre più profonda nella nostra società. Ciò, per problemi che sono complessi, sia dal punto di vista dell'indagine del problema stesso, che dal punto di vista della capacità di rilevarli,

era ciclica. Ogni malattia di questo tipo, che interessa la persona umana, ha una componente personale, psicologica profonda, e ha bisogno dell'apporto sia della farmacoterapia sia della psicoterapia. si sa infatti fino a che punto la malattia può essere indotta da fenomeni ereditari o biologici e fino a che punto viene invece indotta da fenomeni psicologici, di alterazione psico-ambientale e sociale.

è molto diffusa e anche molto difficile da diagnosticare. Talvolta è così oscura anche a se stessi che la persona non vuole ammettere di essere depressa o, se lo ammette, si vergogna di esserlo;

una forte necessità di cambiamento culturale di approccio a questa patologia. È stato detto che la depressione è una malattia come le altre. Io sono un neurologo posso dire che non è una malattia come le altre; posso dire che oggi la depressione, in questo suo modo oscuro di presentarsi, è quasi una patologia sociale, una patologia che sta dentro la nostra società. Non vi è solo la patologia psicotica depressiva, quella che conduce al suicidio, ma c'è la difficoltà di adattamento ai ritmi di questa società, il malessere quotidiano, quello che ha portato

non solo con psicofarmaci ma con droghe e alcool. L'idea che la ricerca della felicità sia tutta chimica francamente è sbagliata; la chimica a nessun livello dà la felicità, né sotto forma di pastiglie per la depressione, né sotto forma di alcool o di altre droghe o sostanze psicotrope. La felicità va ricercata quindi in un modello nuovo di società. Sono convinto che, se si ricercasse un modello più sereno di convivenza, gran parte della patologia depressiva che oggi conosciamo scomparirebbe e con essa anche il consumo smodato e inadeguato di farmaci ansiolitici ed antidepressivi. La mozione

- non si possono trovare in paradisi artificiali. Allora servono centri diagnostici più ampi, che non siano dentro la psichiatria, che vanno costituiti; va costituita una rete per la per la diagnosi e la cura della depressione ed è importante che ci siano anche gli psicologi. Come ho detto, la terapia farmacologica è assolutamente insufficiente, occorre anche un supporto e serve veramente un cambio di marcia più generale nella nostra società.

Chi di noi non ha avuto la tentazione qualche volta di prendere un farmaco ansiolitico, o magari ha avuto momenti di difficoltà e prende un farmaco antidepressivo? Non sapeva a chi rivolgersi, non c'è un centro adeguato se non il centro d'igiene mentale. Non vanno bene i centri d'igiene mentale per curare la depressione così

più relazionali con la gente, in modo che chi ne avverte il bisogno possa avere un riferimento senza necessariamente sentirsi malato o senza dover ricorrere d'altro canto autonomamente ad autoterapie che possono essere assolutamente lesive di sé e

sempre un punto interrogativo subito dopo la parola patologia) per calarla in un momento di socialità delicata, importante e sofferente. La depressione è un è un calvario nel vero senso della parola. È una *via crucis* che non si sa da quale stazione comincia. È un percorso davvero lungo, nell'ambito del quale probabilmente dobbiamo intervenire maggiormente, con una organizzazione sociale importante.

ma soprattutto una percezione umana di contatto con situazioni che si sviluppano nel nascosto della famiglia, nei segreti di una dispersione scolastica che talvolta ci sfugge,

ciò? Vuol dire che ci imbattiamo in una serie di difficoltà dove le solitudini predominano. La depressione è sempre e comunque un momento di solitudine: o una solitudine cercata in uno strano percorso, e in questi giorni stanno venendo fuori

Ricordiamoci che la depressione non è il punto di arrivo di una patologia, sebbene a qualcuno lo possa sembrare. È il dato conclamato di un disagio precedente, ma di frequente è il punto di partenza di un disagio che diviene sempre più drammatico,

i Paesi socialmente più organizzati o quelli meno organizzati? Quelli più avanzati, industrializzati o quelli più arretrati? Se è connesso ad uno stato di povertà, dovremmo trovarlo maggiormente tra coloro che vivono "in depressione economica". Non è così. È veramente un mondo così frastagliato nelle sensibilità quello determinato da queste componenti, nel quale ci si deve interrogare su come vivere in questa società - noi parliamo dell'Italia - in modo ottimale. Occorre una situazione di vita che ci protegga da questo gravissimo sbocco.

le osservazioni formulate dalla collega Sbarbati per quanto riguarda soprattutto il mondo adolescenziale e giovanile, volte a far inserire nelle premesse il punto che evidenzia e che fotografa meglio la realtà, e

Signor Presidente, la problematica delineata nella mozione pone alla nostra attenzione uno dei problemi forse più gravi del nostro Paese, che è all'attenzione del Governo. di una questione di poco conto, considerato che il 18 per cento della popolazione italiana ha sofferto di una malattia mentale nel corso della vita e il 7,3 per cento solo nell'ultimo anno.

cento. Gli impegni che si chiedono al Governo rappresentano certamente uno sviluppo delle attività che il Ministero della salute già pone in essere; c'è però necessità di ulteriori attività, anzitutto a livello centrale, là dove si chiedono azioni di sensibilizzazione della popolazione e di lotta allo stigma,

Signor Presidente, il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia condivide le proposte delineate nella mozione, sia nelle premesse che negli impegni che si chiedono al Governo, alla luce di quanto è stato ulteriormente sottolineato nel corso degli interventi da parte della

In questa breve dichiarazione di voto voglio però dire che tutto questo probabilmente non basta, perché va detto che la perdita costante di punti di riferimento - dalla famiglia all'etica,

un mondo del lavoro sempre più caratterizzato dalla precarietà (soprattutto per i giovani) - e la perdita dei valori di riferimento, che, non dimentichiamolo, hanno accompagnato e tanto hanno contributo allo sviluppo del nostro Paese nel dopoguerra, sono le cause di fondo dell'esplosione di questa patologia. A queste cause se ne aggiunge in questo momento un'altra che abbiamo sottolineato nel corso dei nostri interventi: si tratta di una causa di carattere contingente, ma ugualmente grave, legata alla crisi economica, ai suoi riflessi negativi sull'occupazione e sulle prospettive

a 35 anni è ancora precario, oppure quando tante donne che hanno brillantemente superato corsi di studio anche complicati rimangono disoccupate,

Questa mozione ha due meriti molto significativi. Il primo è il riconoscimento è il riconoscimento di una malattia importante, che colpisce milioni di italiani (come è stato ricordato da tutti i colleghi che mi hanno preceduto), e quindi della necessità della necessità che questa patologia venga inserita nell'integrazione sociosanitaria dei livelli essenziali di assistenza.

da inutili ipocrisie, sappiamo bene che spesso, nei piani di rientro dei deficit sanitari, che ben cinque Regioni importanti del nostro Paese sono state chiamate ad affrontare, i primi servizi, i primi posti letto, i primi presidi di assistenza sanitaria che saltano sono quelli a tutela della salute mentale. ieri la notizia che al Policlinico Umberto I di Roma salteranno i posti letto di assistenza a due importanti patologie, l'anoressia, che tra l'altro è una delle maggiori cause di mortalità della popolazione giovanile femminile,

per la vita sociale del nostro Paese, per le conseguenze sulla qualità della vita dei nostri concittadini, sulla efficienza ed efficacia con cui essi possono assolvere alle loro funzioni e alla loro attività lavorativa. Addirittura, vi è un interessante e importante studio dell'Organizzazione mondiale della sanità che quantifica, con calcoli e con formule matematiche, il costo sociale della patologia depressiva, pari a quello che possono determinare le patologie coronariche e l'infarto miocardico acuto e, addirittura, al doppio delle patologie neoplastiche. In tal modo, possiamo renderci conto di cosa stiamo discutendo.

Si tratta di una patologia sottodiagnosticata e, quindi, vi è la necessità di informare e di formare. È una patologia maltrattata e, quindi, vi è la necessità di parlare di qualità e di appropriatezza dei servizi. È una patologia che non ha alcuna sussidiarietà nei servizi sanitari del nostro Paese, perché manca il necessario collegamento tra medicina di base, che è la prima trincea alla quale si rivolge il cittadino, i centri di salute mentale e i distretti sanitari di base. Questa mozione, nella sua semplicità, tocca e dà al Governo un impegno su tre direttrici: la sensibilizzazione, l'appropriatezza delle prestazioni (perché l'uso e l'abuso di farmaci, che i colleghi Bosone e Saccomanno hanno messo in risalto, determinano anch'essi un'elevazione dei costi della politica sanitaria)

d'integrazione anche in questo settore così importante e delicato, portano a far sì che il piano nazionale di prevenzione

mondo della patologia medico-sanitaria come uno degli obiettivi da perseguire. Anche questo non è pacifico,

lo dico al rappresentante del Governo: su questo piano lo Stato ha impegnato 200 milioni di euro di fondi, ma mancano due aspetti. Il primo è un monitoraggio e un controllo sul modo in cui vengono spese queste risorse dalle singole Regioni. Il secondo aspetto consiste nella necessità di eliminare sempre di più una disuguaglianza territoriale e sociale esistente all'interno del nostro Paese.

la buona politica si deve dare: che questa mozione non crei soltanto l'illusione di avere parlato del problema, di essere tutti con la coscienza a posto. posto. La politica che crea illusione, infatti, crea successivamente delusione, e la delusione, signor Sottosegretario, è l'anticamera

tratta di una mozione condivisibile e molto attuale. Non dobbiamo sottovalutare che nella previsione fatta dall'Organizzazione mondiale della sanità la depressione costituirà nel 2020 la seconda causa di disabilità nel mondo e la prima causa per quanto riguarda le donne.

concetti già espressi nel dibattito di questa mattina, che è stato particolarmente costruttivo. In realtà, è emerso molto chiaramente che il problema esiste e ha una gravità sconvolgente. Rinvio alle parole della presentatrice della mozione, la senatrice Baio, per quanto riguarda i possibili drammatici risvolti di questa patologia, fosse anche solo - permettetemi, il "solo" - in tema di suicidio, con i numeri che abbiamo appena

in maniera estremamente chiara che il Governo dà un parere favorevole a questa mozione e che dal punto di vista tecnico il Ministero si sta già muovendo per dare risposte in questa direzione; ma la preoccupazione che ha espresso il sottosegretario Caliendo è ovviamente quella che pervade

Ebbene, gli strumenti secondo me ci sono. Rimanendo in tema di depressione, a firma mia e della collega Boldi, ad esempio, è stato depositato in data 4 marzo 2009 un disegno di legge intitolato «Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e disposizioni in materia di tutela della salute mentale» che potrebbe sembrare un disegno di legge megagalattico che vuole andare a soppiantare completamente la legge n. 833. In realtà, non è assolutamente così. È un disegno di legge estremamente specifico, che ha come punto punto centrale proprio la terapia della depressione nella sua metodologia di sviluppo sul territorio, andando a separare nettamente le strade

Dietro a questa definizione, vi è problema di fondo non indifferente, e cioè, che mentre le patologie psichiatriche unanimemente conosciute

a cui i pazienti, affetti da questo dramma, possano afferire. I costi ai quali la senatrice Baio e gli altri colleghi negli interventi che si sono susseguiti facevano riferimento non sono i costi reali della terapia psichiatrica, ma sono quelli indotti dalla mancata terapia della patologia psichiatrica. Credo che questo sia il punto saliente su cui dibattere;

un presidio di trattamento della patologia psichiatrica - infatti, nel momento in cui la patologia insorge è assolutamente curabile con risorse assolutamente limitate andremmo a risparmiare decine di migliaia di milioni di euro dal bilancio. Una volta tanto inoltre un disegno di legge non avrebbe bisogno di coperture economiche ma determinerebbe un risparmio dal punto di vista economico, semplicemente separando le due linee di finanziamento tra la cosiddetta patologia psichiatrica nobile rispetto a questa assolutamente più subdola.

La senatrice Bianchi ha depositato un disegno di legge *ad hoc* per questo, al quale chiedo ora di poter aggiungere la mia firma. Ma chiedo anche, non tanto al Governo ma al Parlamento, di prendere le risorse già esistenti in Parlamento per combattere questo tipo di patologia in modo da non limitarci alla mozione, che è un impegno banale, ma fare qualcosa davvero di concreto. E qui ringrazio il senatore Mascitelli che ci stimola a non avere le illusioni ma a fare qualcosa di concreto. Io credo che qualcosa di concreto sia assolutamente la mozione è condivisa; i disegni di legge potrebbero essere assolutamente condivisi; i problemi della copertura economica potrebbero essere assolutamente superati e superabili. Potrebbe essere la volta che da una mozione nasca davvero un disegno di legge condiviso che vada a risolvere davvero un grande problema, dando una risposta concreta ad un problema reale di questo Paese che - ripeto ancora - è assolutamente misconosciuto ma presenta risvolti a dir poco drammatici.

Signor Presidente, il nostro voto sarà convintamente a favore della mozione presentata dalla senatrice Baio, che raccoglie consensi *bipartisan* in questa Aula. La ringraziamo per questa iniziativa che ci ha consentito oggi qui di discutere e di approfondire tale questione, di creare anche una cultura politica, il che non è indifferente in tempi come questi, e di spronare il Governo a trovare delle risposte e delle soluzioni per affrontare questa

purtroppo, anche i bambini, e sempre di più gli adolescenti, come è stato ricordato, e in particolare colpisce le donne. Su questo vorrei brevemente soffermarmi, perché in molti degli interventi è stata sottolineata, questa particolare predisposizione delle donne che, nella loro vita, attraversano dei momenti particolarmente complessi, come quelli della gravidanza, del parto e del climaterio,

solitudine queste fasi, addirittura affrontando le difficoltà del mondo del lavoro che le respinge proprio in questo momento e che cerca di espellerle dal processo produttivo. vivono questa difficoltà perché le famiglie, sempre più piccole numericamente, non sono in grado di dare loro sostegno in momenti importanti come quello della gestazione e della nascita di una nuova vita. Addirittura gli ospedali hanno ridotto così tanto i tempi di degenza che la donna che partorisce non riesce a riprendersi, se non dalla fatica psichica, nemmeno dalla fatica fisica del parto.

all'insorgere di depressioni *post partum* che alcune volte non vengono curate e, quindi, sfociano nelle situazioni drammatiche che la cronaca quotidiana ci riporta; ci ricordiamo di questo problema ed alziamo alti lamenti, ma finito il momento dell'emozione non succede assolutamente nulla: i nostri consultori sono sempre più ridotti al lumicino e non c'è più un'assistenza territoriale in grado di supportare questo problema. Anche quelle donne, quindi, che se la cavano abbastanza bene,

vita. Nel rapporto dell'ONU «Donne nel mondo 2010», che è stato presentato il 28 ottobre scorso, si sottolinea un fatto importante, cioè che nel mondo le donne hanno fatto dei grandi passi in avanti sia sul piano dell'istruzione, sia su quello della cura della propria salute, ma rimane un forte ed evidente *gap* di genere nella vita familiare, pubblica e politica che è appesantito anche dalle discriminazioni e dalle violenze e che è difficile colmare. Quindi, le donne subiscono discriminazioni nel mondo del lavoro,

grava la gran parte dell'impegno nelle attività di cura dei bambini e degli anziani e nelle attività domestiche, anche quando lavorano fuori casa. Nessuno si è chiesto quanto ciò comporti, di fatto, una forte sensazione di inadeguatezza da parte delle donne che sostengono tale enorme carico di lavoro durante la loro vita produttiva. Questo porta stanchezza, porta appunto al senso di depressione; è un veicolo verso la depressione. A ciò poi si aggiungono, purtroppo, i casi di violenze e maltrattamenti all'interno delle pareti domestiche che qui sono stati ricordati, difficili da individuare e superare. Sono condizioni che, protratte nel tempo, portano a vivere in uno stato di paura e di annullamento di sé,

che la lotta alla depressione venga costruita non solo sul piano dei servizi sanitari, ma con una strategia più ampia di carattere più generale, trasversale. Abbiamo diversi Ministeri che si potrebbero occupare di questo tema per favorire il superamento delle condizioni che dicevo prima, che sono poi portatrici di tale malattia. Entrando nel merito delle proposte fatte, è chiaro che

chiedere nuovi servizi, in una condizione in cui si tagliano quelli esistenti, diventa abbastanza difficile. Il senatore Mascitelli ricordava il caso del Policlinico Umberto I di Roma, grande centro di cura e ricerca di interesse nazionale, se non anche sovranazionale,

delle assunzioni del personale, per cui chi lavora in quel reparto è costretto a fare l'impossibile per mantenere funzionante un servizio che non ha soltanto una funzione di cura nell'ambito ospedaliero, ma si rapporta al territorio per la cura dei casi che gli sono proposti. È pertanto chiaro che di fronte a tale situazione diventa difficile poter proporre nuovi interventi. Credo però che, visto che si è fatto il piano socio-sanitario nazionale e che lo stesso è stato concordato, senza che naturalmente noi ne potessimo in qualche modo discutere, con le Regioni, sarebbe interessante sapere quali sono le priorità, gli obiettivi-salute che ci poniamo in questo Paese. Anche rimanendo nell'ambito Paese. Anche rimanendo nell'ambito delle risorse esistenti, credo infatti che, se si definissero quali sono gli obiettivi-salute,

che cosa osta a dire che parte delle nostre risorse devono poter essere indirizzate in questa direzione, magari razionalizzandone altre che oggi per le patologie ricorrenti non ricorrenti non sono necessarie? Ecco, non siamo qui per dire che bisogna espandere la spesa, perché sappiamo che in questo momento sarebbe solo un atto propagandistico. Siamo a chiedere che si riordini la spesa sanitaria secondo obiettivi-salute condivisi, come quello che abbiamo condiviso oggi in quest'Aula.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghe e colleghi, siamo tutti d'accordo nel riconoscere come la depressione sia una patologia dell'umore con sintomi comportamentali, somatici e affettivi che possono gravemente diminuire la personalità, nonché la capacità del depresso di adattarsi alla vita sociale. È stato ricordato come l'Organizzazione mondiale della sanità metta la depressione attualmente al quarto posto nella graduatoria delle disabilità e come questa tendenza crescerà nel 2020. La scienza ha ormai confermato che la depressione non ha soltanto origini psicologiche, ma anche biologiche e coinvolge specifici sistemi neurotrasmettitori per la serotonina, la dopamina e la noradrenalina. Il depresso, se curato, nel 75 per cento dei casi può guarire o avere comunque una condizione di vita migliore per se stesso e per i familiari, che spesso non riconoscono la gravità il dramma esistenziale del malato congiunto. ci chiediamo come si sia potuti arrivare a questo, perché non sia stato capito, perché la persona non sia stata curata, e siccome stiamo parlando di una patologia curabile, dobbiamo riconoscere che si deve procedere con un piano personalizzato nella terapia, sia psicologico che farmacologico. Infatti, gli antidepressivi non sono tutti adatti a un protocollo generale, ma devono essere adattati a ogni singola persona. Trovo molto importante la nostra discussione di oggi, ma soprattutto è importante la sensibilizzazione di massa perché la depressione venga riconosciuta e considerata come una malattia curabile, promuovendo anche iniziative per sostenere la persona depressa ed aiutarla a rivolgersi ad un medico specialista. Per tutto questo non credo ci debbano essere risorse ulteriori. Si parla dei cosiddetti tagli dei cosiddetti tagli alla sanità, ma non mi sembra che in Italia, in molte Regioni, anche in momenti in cui le risorse erano maggiori rispetto ad oggi, si sia fatto molto per uniformare o garantire a tutti l'accesso alle cure. Credo che il problema vero sia quello dell'organizzazione e dello sfruttamento delle risorse che si hanno: in questo caso, a proposito della depressione, i medici di base, che devono essere sensibilizzati; i consultori familiari, che devono ritornare ad essere potenziati con il personale esistente e a svolgere il ruolo che era nell'intenzione nel momento in cui sono stati creati. Il consultorio familiare deve essere vicino alla famiglia

può e deve essere una riorganizzazione di questa rete, si possono individuare percorsi terapeutici anche al di fuori dei consueti. Non sono d'accordo, ad esempio, quando si grida all'allarme sui posti letto tagliati per i pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare. che personalmente ne sono quasi felice; infatti, le persone affette da disturbi del comportamento alimentare attualmente sono ricoverate in repartini psichiatrici ed è una cosa abominevole, perché dovrebbero essere

Si potrebbe certamente opinare sul passaggio diretto dal Governo alla commissione da parte di un esponente prestigioso come il Vice Ministro, ma ben altri sono stati i passaggi scandalosi, dalle banche alla CONSOB e viceversa, che hanno configurato rapporti incestuosi, come nel caso del signor Vittorio Conti, proveniente da Banca Intesa, o degli ultimi due direttori dell'ABI, Giuseppe Zadra e Giovanni Sabatini, provenienti dalla CONSOB, in un consolidato sistema di porte girevoli che ha provocato, per omessa vigilanza, una lunghissima catena di crack finanziari ed industriali che hanno ridotto sul lastrico un milione di risparmiatori, per un controvalore di 50 miliardi di euro. Ho sempre chiesto dove erano

ad un sepolcro imbiancato iniziando a fare piazza pulita di quei dirigenti, che invece di sanzionare i derivati avariati delle banche e di Unicredit hanno inseguito teoremi con l'unica finalità di intimidire e ricattare quei rappresentanti dei risparmiatori che difendono i diritti di tanta povera gente truffata dalle banche. Quindi, ci auguriamo che il presidente Vegas possa rappresentare un fattore di discontinuità per ridare prestigio a un'autorità che